Comunico che, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la seduta costitutiva della Commissione parlamentare per la semplificazione, già prevista per oggi, è rinviata a martedì 26 marzo 2024, alle ore 14, presso la sede di Palazzo San Macuto.

sociali*. Signor Presidente, signori senatori, vi è l'urgenza nel nostro Paese di implementare la cultura della sicurezza in tutti gli ambiti della vita lavorativa. Mai avrei voluto assistere a nuove tragedie sul lavoro. Ciononostante, siamo costretti ad affrontare questo tema, non senza aver prima rivolto un pensiero alle vittime e alle loro famiglie.

Con la presente informativa intendo condividere gli interventi e le azioni più recenti che il Governo ha posto in essere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I fatti accaduti di recente a Firenze e le tragedie che ci troviamo ad affrontare troppo spesso, quasi quotidianamente, ci costringono a confrontarci con una realtà che necessita non solo di interventi ben definiti, ma anche di una nuova cultura e consapevolezza della tutela della salute e della sicurezza. Solo qualche mese fa, in questa stessa Aula, la convergenza tra maggioranza e opposizione su un tema così delicato, da essere comune a tutte le forze politiche, ha permesso l'approvazione di una mozione unitaria che impegnava il Governo a mettere in campo una serie di azioni. Oggi, nel mio ruolo di Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rendo questa informativa per darvi conto di quanto fatto anche rispetto agli impegni presi. Fin dal nostro insediamento, il Governo è intervenuto al fine di arginare il fenomeno delle morti bianche e dei gravi infortuni sul lavoro. Lo abbiamo fatto pensando non solo ai lavoratori di oggi, ma anche a quelli di domani, con interventi trasversali che guardano al mondo del lavoro, delle imprese e della scuola e improntati alla prevenzione e alla formazione, alla sensibilizzazione e alle azioni concrete di contrasto all'irregolarità. azioni urgenti e doverose, non da ultimo per dare un segnale forte a quei datori di lavoro che pensano di poter eludere il sistema delle regole a tutela dei lavoratori e anche agli stessi lavoratori che devono contribuire a far implementare la cultura della sicurezza in ambito lavorativo. Posso dire che, rispetto ai punti della mozione approvata a settembre, molti interventi erano già in corso di definizione e altri sono stati coperti dai più recenti provvedimenti non governativi. Il provvedimento normativo che è all'esame delle Commissioni della Camera dei deputati in questi giorni - il decreto-legge 2 marzo 2024, risponde proprio a queste esigenze e contiene un pacchetto di norme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recanti disposizioni in materia di contrasto al lavoro sommerso e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Su queste disposizioni normative è in atto un confronto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e datoriali sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza. Con riferimento agli interventi effettuati nel decreto-legge PNRR-*bis*, abbiamo anche avuto modo di confrontarci con le parti sociali e datoriali e abbiamo insediato un tavolo che si riunirà a cadenza settimanale per accompagnare l'implementazione delle norme, con un primo intervento tenutosi il 15 marzo scorso, poi successivamente il 18 marzo e, infine, è già programmata una riunione per il prossimo 26 marzo. Si tratta di un confronto concreto sulle disposizioni per mantenere aperto un dialogo fattivo e costante con le parti sociali e datoriali e raggiungere insieme l'obiettivo di un più effettivo contrasto agli infortuni nei nei luoghi di lavoro. Passando al merito dell'intervento normativo, rilevo che abbiamo provveduto al potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questo è il Governo che più di tutti ha rafforzato il numero e gli strumenti a disposizione degli ispettori del lavoro. Tra quelli che abbiamo già assunto e quelli previsti dalle nuove norme, ai 2.300 che avevamo in servizio ne aggiungiamo oltre 1.600. Di questi ultimi, circa 800 ispettori tecnici sono già stati assunti e sono già in servizio. Con le più recenti disposizioni, abbiamo prorogato sino al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni all'assunzione di personale ispettivo non utilizzate dall'Ispettorato nazionale

in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e di 50 unità di personale per l'Arma dei carabinieri. A questo si deve aggiungere l'intervento che abbiamo fatto

L'INL avrà inoltre la possibilità di bandire concorsi su base regionale, così da garantire una copertura maggiore dei posti vacanti, oltre a poter contare su un rafforzamento del trattamento economico complessivo; ciò al fine di scongiurare ciò che è accaduto nel recente passato, ove molto spesso i vincitori di concorsi hanno deciso di rinunciare all'impiego a causa della lontananza dalla sede e del trattamento retributivo. In questo modo, l'obiettivo del Governo è mettere a disposizione dell'Ispettorato un contingente ancora più ampio di personale tecnico addetto al controllo dei luoghi di lavoro. A A questo proposito, rilevo che nel 2023 abbiamo avuto un incremento del 20 per cento delle ispezioni, che arriverà anche grazie al completamento della formazione del personale, assunto lo scorso anno, al 40 per cento nel 2024. Quando avremo in servizio l'intero contingente per cui abbiamo legiferato, avremo la possibilità di raddoppiare la nostra forza e, quindi, il numero delle ispezioni che potranno essere messe in campo. Con la mozione di cui parliamo ci eravamo impegnati a effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto e il distacco da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza

al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, sia sul piano penale con la reintroduzione e l'aggravamento delle sanzioni penali di contrasto al fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Siamo inoltre intervenuti in tema di appalto fittizio con l'estensione della responsabilità solidale tra committente, imprenditore o datore di lavoro e appaltatore o subappaltatore nei confronti dei lavoratori anche alla figura dell'appaltatore fittizio, ovvero di colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. In questo modo, mentre oggi l'appaltatore fittizio non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro, non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative, da questo momento sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto. Sempre nell'ambito degli appalti pubblici e privati, secondo le nuove disposizioni il responsabile unico del procedimento (RUP) o il committente dovrà richiedere il certificato di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. Ferme restando le soglie e le responsabilità già previste dall'apposito decreto ministeriale, che disciplina la congruità del costo della manodopera e i relativi oneri per le imprese edili esecutrici dei lavori, la nuova disposizione introduce una specifica sanzione, colpendo gli autori delle condotte di natura omissiva. Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell'azienda e di favorire nel contempo l'emersione del lavoro irregolare, è stata prevista una disciplina specifica in materia di *compliance*. In caso di pagamento spontaneo effettuato entro un certo termine, vengono ridotte le sole sanzioni sole sanzioni previste dalla normativa vigente - lo sottolineo - e vi è la possibilità di accedere al cosiddetto ravvedimento operoso, nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente da parte del datore di lavoro prima della contestazione o della richiesta da parte dell'ente impositore. A settembre ci eravamo impegnati a introdurre disposizioni in favore delle imprese che assicurassero ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendessero responsabili di violazioni in tema di sicurezza. Abbiamo rispettato entrambi gli impegni. Da un lato, con la lista di conformità dell'INL, introduciamo uno strumento in favore dei datori di lavoro che dimostrino comportamenti corretti e rispettosi delle regole nella gestione dei rapporti di lavoro. I datori di lavoro che siano stati oggetto di accertamento ispettivo, da cui non sia emersa alcuna violazione o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, saranno iscritti nella lista di conformità, che è un apposito elenco informatico informatico consultabile pubblicamente. L'iscrizione alla lista di conformità dell'INL determina la mancata sottoposizione, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, a ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti. Resta la possibilità di effettuare verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche a seguito di specifiche richieste di intervento, nonché di indagini demandate dalle competenti procure della Repubblica. Dall'altro lato, dopo sedici anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, introduciamo un sistema di qualificazione delle imprese, la cosiddetta patente a crediti, che i sindacati e diverse forze politiche chiedevano da anni, agendo per una maggiore responsabilizzazione delle imprese. La patente costituirà, a decorrere dal 1° ottobre 2024, un titolo abilitativo il cui possesso consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nell'ambito di cantieri temporanei o mobili. Nell'elaborare questo strumento, due sono stati i principi ispiratori: la sicurezza e la formazione. Perciò, se la patente subisce una decurtazione dei punti a seguito di violazioni in materia di salute e sicurezza, deve rilevarsi che proprio la formazione in quelle stesse materie consente il riacquisto dei crediti perduti. Il garantismo fa sì che le decurtazioni avvengano solo qualora siano stati adottati provvedimenti definitivi, definitivi, sanzionatori o di accertamento. Questa è una norma dello Stato e un principio assolutamente da ricordare. Tuttavia, per rendere efficace lo strumento, abbiamo previsto che nelle ipotesi più gravi, ovverosia nei casi in cui si sia verificata la morte o un'inabilità un'inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, valutate le circostanze del caso concreto, abbia facoltà di sospendere in via cautelativa la patente fino a un massimo di dodici mesi. Garantire maggiore consapevolezza, ma anche una formazione costante e ulteriore rispetto a quanto già ampiamente previsto dall'apposito Testo unico sulla sicurezza, è il principio che contraddistingue le previsioni in materia di riaccreditamento della patente. Dunque, per rafforzarne la valenza e l'importanza, abbiamo previsto l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verifica del possesso della patente non solo nei confronti dell'impresa affidataria, ma in generale di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi presenti sul cantiere, anche e soprattutto in virtù di subappalti. Questo al fine di responsabilizzare tutti i soggetti che a diverso titolo intervengono sui cantieri e hanno poteri e obblighi nei confronti dei lavoratori. Vorrei sottolineare che la patente è stata definita a crediti, perché ovviamente non mira ad attribuire un punteggio alla vita umana, che ha un valore incalcolabile su cui credo non si debba ironizzare, o ad altri infortuni che possono riguardare i lavoratori, ma mira a qualificare le imprese come strumento di riconoscimento di quelle virtuose che operano correttamente sul mercato. anche rispetto agli impegni relativi alla promozione della cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento a ogni livello di istruzione e formazione, prevedendo altresì il coinvolgimento con apposite attività formative delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento *ad hoc*. La consapevolezza dei propri diritti e doveri, soprattutto in ambito lavoristico e di sicurezza, è un valore che dobbiamo trasmettere ai più giovani. Gli studenti di oggi saranno i lavoratori e i datori di lavoro di domani e devono essere coscienti di quanto le loro azioni possano incidere su di sé e sugli altri. Tocca a noi come adulti, ma soprattutto come rappresentanti delle istituzioni, dotarli di tutti gli strumenti necessari per responsabilizzarli già da oggi. Diverse sono le iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che sono rivolte ai giovani e che vedono una capillare ed estesa rete di collaborazioni interattive e sinergiche con diversi soggetti istituzionali, che ha consentito e consente tuttora di condividere strategie finalizzate ad adottare politiche attive in materia di salute e sicurezza. Mi piace citare, tra le diverse iniziative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il bando di concorso nazionale dal titolo «Salute e sicurezza insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola», indetto d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito. Ho accolto con favore l'approvazione alla Camera della proposta di legge che introduce l'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far acquisire le conoscenze dei capisaldi dell'ordinamento e delle principali normative che riguardano il lavoro. Le finalità perseguite sono comuni al percorso del nostro Esecutivo e sono connesse alla necessità di contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore, affinché siano responsabili e attivi nel rispetto delle regole connesse a questo *status.* Il coinvolgimento delle vittime stesse di infortuni che portino la loro testimonianza potrà stimolare una riflessione sulla rilevanza della materia e divulgare maggiormente e in modo migliore l'importante messaggio del valore della prevenzione in grado di investire ogni aspetto della vita quotidiana.

prevedendo per l'anno scolastico accademico 2023-2024 l'estensione della tutela assicurativa INAIL allo svolgimento delle attività d'insegnamento e apprendimento

Non solo: in quell'occasione avevamo anche istituito il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. In merito alle nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, per il rafforzamento delle tecniche degli istituti di prevenzione e il miglioramento dell'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio, ricordo che è stato istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), diretto a orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Sono stati avviati i lavori per la sottoscrizione di una convenzione quadro che ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le parti firmatarie (INAIL, Regioni e Province autonome) per l'accesso e l'utilizzo a titolo gratuito dei servizi del SINP denominati flussi informativi, registro esposizione e cruscotto infortuni. La Convenzione è stata firmata il 20 novembre 2023 dal commissario straordinario dell'INAIL e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. che, nel bilancio di previsione 2024 dell'INAIL, sono raddoppiate, rispetto al 2023, le risorse impiegate per le politiche di prevenzione in materia di sicurezza.

a promuovere la riduzione del fenomeno infortunistico. Altrettanto importante è l'investimento in formazione, destinato alla crescita delle competenze dei lavoratori e degli operatori della sicurezza, che da oltre 10 milioni passa a 50 milioni di euro. I 508 milioni di euro rappresentano l'importo più alto stanziato nelle quattordici edizioni dell'iniziativa del bando ISI. Sono inoltre aumentate a 200 milioni le risorse per la riduzione del premio assicurativo delle imprese che realizzano interventi migliorativi per la prevenzione. Inoltre, è nostra intenzione raddoppiare, portandolo a 800 milioni, lo stanziamento per il *bonus* riservato alle aziende che registrano un calo di infortuni e malattie: un incremento che determinerebbe un investimento annuale complessivo per la sicurezza superiore a 1,5 miliardi di euro. Siamo tutti consapevoli che la strada è ancora lunga. L'obiettivo che tutti ci prefiggiamo è di arrivare, in un tempo non lontano, ad avere un numero di incidenti e di vittime sul lavoro pari allo come ho fatto già in occasione della riunione tenutasi con le organizzazioni sindacali e datoriali la scorsa settimana, il primo di una serie di incontri di carattere tecnico, come vi dicevo - chiamo tutti alla responsabilità e alla collaborazione. Come fatto in occasione della mozione approvata a settembre, dobbiamo proseguire sulla strada della collaborazione per ottenere importanti risultati per i lavoratori e le loro famiglie. Quanto abbiamo fatto è un passo importante, da cui non intendiamo tornare indietro. Ma siamo consapevoli che tutto sia perfettibile e, pertanto, siamo disponibili a confrontarci sulla base di proposte e idee concrete in grado di migliorare la qualità della vita dei lavoratori e preservarne l'integrità. la ringrazio per la sua informativa su un argomento che sta veramente a cuore a tutti i Gruppi del Senato.

come il presidente La Russa ci ricordava - riscontra una sensibilità trasversale che riguarda tutte le forze politiche, per cui ciascuno di noi è tenuto a tenere toni conformi alla gravità di ciò di cui stiamo parlando. Purtroppo, stiamo parlando di una strage continua che - secondo i dati ufficiali

ma a volte le dimensioni del fenomeno rischiano di essere anche maggiori di quelle contabilizzate. Giustamente, ci siamo alzati tutti nel ricordare i morti sui luoghi di lavoro. Questa mattina, alle ore 8, a Lucca, è morto un uomo di cinquantadue anni, caduto all'interno dello scavo di un cantiere stradale.

Non parliamo più dunque di morti bianche, né di fatalità. Cerchiamo di affrontare una guerra che ogni giorno dobbiamo fronteggiare e che purtroppo riguarda la responsabilità di tutti i Governi. Lei ha citato il tema del PNRR e delle disposizioni sulla patente a punti. Condivido con lei l'idea che la vita umana non possa avere un punteggio

Signor Ministro, lei ha detto che c'è stato un aumento di ispettori del lavoro di oltre 1.600 unità, tra quelli già in organico e quelli che vi entreranno. Condivido l'idea di investire sulle persone dell'Ispettorato del lavoro, ma lei sa meglio di me che, se le persone che devono effettuare i controlli non hanno gli strumenti per farli, il rischio è che poi al numero effettivo di persone che entrano non corrisponda un'efficacia nei controlli e nelle sanzioni.

Signor Ministro, dei 7,2 miliardi assegnati al Ministero del lavoro sono stati spesi solo 59 milioni di euro, meno dell'1

un altro punto. Signor Ministro, introduciamo una *sandbox* regolamentare sul lavoro. So che questo tema coglie la sua sensibilità: utilizzare gli strumenti della transizione digitale, in particolare

non hanno i *database* per utilizzare, attraverso algoritmi di intelligenza artificiale generativa, gli investimenti sulla prevenzione e sulla sicurezza, rischiamo di non dar loro gli strumenti per

del *vulnus* più grande che può capitare alle persone e a un popolo, quello di coniugare il diritto più importante che abbiamo oltre a quello alla serenità, quello al lavoro, che però produce vittime, non si può essere mai felici, casomai sereni.

di colmare il più possibile questa contraddizione che urta contro la democrazia, il diritto, la serenità che il lavoro dà e le vittime

causano. Come abbiamo detto ieri, parlando di Ilaria Alpi, in questa benedetta - qualche volta, maledetta - primavera, dove c'è oscurità,

nell'attività lavorativa, anche quella regolare, regolamentata da leggi e procedure apparentemente positive. però per la fretta, per l'ingordigia o per la voglia di ottenere tutto, subito e troppo, si patteggia con la vita delle persone più indifese. È veramente insopportabile, per che un genitore esca da casa e non vi torni più. Questo clima di incertezza offende e ferisce. Credo quindi che il suo provvedimento e l'attenzione del Governo a questo tema siano un passo in avanti positivo importante, anche se - come lei ha detto bene - non decisivo, perché si può e si deve sempre migliorare. Signor Presidente, questa mattina sono molto lieto anche di essere vicino al presidente Zaffini, perché insieme abbiamo fornito al ministro per le disabilità Locatelli un nuovo strumento di valutazione dell'invalidità, del quale il lavoro e

come condizionato: sì, lo sono dal bene comune, dall'affetto che mi dà stare qui e anche dalla positività della lotta in difesa delle disabilità

dicendo che esiste anche una forma di nocività lavorativa (e anche di morte, soprattutto psicologica) per centinaia di migliaia di persone con disabilità,

ma si può anche morire dentro, autocensurandosi, perché sembra che la società non dia risposte alla voglia di integrazione lavorativa di tante persone con disabilità.

per affrontare organicamente la questione, e lo ha fatto scevra da ragionamenti politici di parte. È la sua cifra, Ministro, ed è la prima occasione nella quale posso riconoscerle questo merito, dal mio punto di vista, che è esaltato dal fatto che oggi stiamo parlando di una questione che riguarda tutti e che deve vedere tutti coinvolti con il massimo della sobrietà e della capacità di interlocuzione con gli altri. Si tratta di una piaga che oggettivamente per il nostro Paese è estremamente grave, per cui plaudo al fatto che il Governo le consenta di lavorare. Se ho un rammarico è che - a mio modo di vedere - personalità come la sua dentro questo Governo non sempre sono messe nella condizione di fare tutto quello che potrebbero.

a cercare di essere più efficaci. L'altra questione, che non è citata nella relazione - a mio avviso - apre tutta una tematica relativa non soltanto all'infortunistica. La relazione infatti

abbastanza sconsolante che fino ad oggi non sia stata messa in campo un'iniziativa che agisca con un occhio rivolto a ciò che è avvenuto nel passato.

legati all'attività petrolifera e alle centrali ENEL. Tutti sappiamo perfettamente di cosa stiamo parlando. Ricordo che il rischio dell'amianto riguarda non soltanto le persone che sono state coinvolte in quei cantieri, ma anche le famiglie che magari hanno visto arrivare a casa le tute da lavoro

efficace anche sui familiari di quelle vittime che magari hanno avuto conseguenze gravissime, con perdita di vite umane? Questo è un primo tema che le sottopongo. Ragioniamo sul tema degli incidenti sui luoghi di lavoro in termini più organici e proviamo a mettere in campo delle iniziative che riguardino anche il tema della salute delle persone e delle famiglie coinvolte. È una proposta che naturalmente deve vedere coinvolto anche il ministro Schillaci e le preannuncio che da parte nostra arriverà probabilmente una proposta di legge su questo punto. Passo all'altra questione.

iniziative del suo stesso Governo, per opera di altri Ministri, che sono andate esattamente nella direzione opposta. Il codice degli appalti di Salvini, con la reintroduzione del massimo ribasso, non è un aiuto a frenare il tema degli incidenti sul luogo di lavoro. così forte sulla questione del PNRR, quello doveva essere un criterio. Chi le parla non la pensa come Lombardo,

Una delle cifre importanti del suo lavoro è stata aver rimesso al centro il tema della partecipazione agli utili e del coinvolgimento dei lavoratori dentro le aziende. Ovviamente a questo si deve

Grazie, Presidente. Il controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro. Perché non istituire delle commissioni aziendali - è una proposta che copio, pari pari, da Oscar Giannino, che secondo me ha fatto un ragionamento giusto - all'interno delle aziende per fare in modo che i lavoratori possano segnalare, sulla base della loro esperienza, criticità come quelle, per esempio, relative ai macchinari che hanno ucciso

Lei li avrebbe approvati, ma alla fine, dentro la sua maggioranza, è prevalsa la volontà di farli ritirare. Quegli emendamenti avrebbero introdotto un blocco a quei macchinari che hanno ucciso quella ragazza e sarebbero oggi estremamente importanti al fine di garantire sicurezza sui luoghi di lavoro.

io sono molto sensibile, ho anche qualche responsabilità e quindi mi sento in colpa per alcune questioni non affrontate. Però voglio intervenire in modo chiaro rispetto alle cose che ho sentito prima,

la Ministra ha spiegato le cose che sono state fatte, le norme che sono state cambiate o che sono in via di cambiamento, ma quello che non funziona, Ministra, è un dato: lei dice di aver coinvolto i sindacati e le parti sociali, ma io registro che alcuni sindacati importanti hanno dichiarato sciopero e associazioni datoriali importanti hanno dichiarato insoddisfazione. Quindi, di fronte a quello che è successo, il dato importante è cambiare le norme, ma il problema principale è costruire - a mio avviso

lavoro precario e subappalti al massimo ribasso hanno portato all'attuale situazione. Tutti gli incidenti plurimi ci squadernano questo fatto.

la presunzione di avere la verità in tasca. Per questa ragione è importante il coinvolgimento dei soggetti, in particolare dei rappresentanti delle imprese e dei rappresentanti dei lavoratori. Se mancano questi elementi, manca sostanzialmente il collante per poter invertire questa tendenza.

non dovrebbe conoscere e non conosce - come ha detto lei - alcun colore politico. È un argomento importante e la ringrazio per il lavoro che sta facendo.

Solo così possiamo evitare nuovi incidenti. Non è più sopportabile - come ha detto qualcuno e come ha sottolineato anche lei - ascoltare sempre annunci di morti sul lavoro. L'idea di non tornare a casa a causa di un incidente sul lavoro che ha portato alla morte, e quindi non poter più vedere i propri affetti, è davvero una cosa insopportabile, ma soprattutto davvero impensabile. Non può esserci attività per la quale si deve o si possa morire. Oltretutto, i morti sul lavoro appartengono quasi sempre a quelle categorie che hanno contratti e ruoli con con retribuzioni molto basse. Questa è anche una condizione molto odiosa, mi permetta: lavorare per una paga modesta per la quale si può morire è intollerabile. L'idea della patente a punti per le imprese, che è stata oggetto di un disegno di legge presentato dal Gruppo Forza Italia qui in Senato, di cui sono prima firmataria - ne sono molto contenta - è stata accolta immediatamente dal Governo.

È giusto che si aumentino i controlli, per cui trovo corretto incrementare il numero degli ispettori del lavoro che possono e devono verificare il rispetto delle regole sulla sicurezza. È bene anche ricordare che il primo controllo deve essere effettuato dai responsabili della sicurezza di ogni azienda, che devono avere il quadro esatto sulle condizioni di salute e di tranquillità dei luoghi dove lavorano ovviamente, stare attenti che non ci siano dei rischi. *In primis* devono essere i lavoratori stessi a denunciare, qualora percepiscano di avere condizioni di non tranquillità. I lavoratori devono essere sempre i primi a poterlo dire e devono fermarsi per non rischiare la loro vita. Bisogna quindi mettere in campo iniziative serie e non solo formali, sempre a tutela dei lavoratori.

al rischio che corrono in quel momento nel luogo di lavoro dove si trovano. Signora Ministra, desidero quindi dirle che l'attività economica e la sicurezza sul lavoro devono diventare sinonimi: questo è un dato molto importante. intervento, l'appoggio di Forza Italia a ogni iniziativa che renda più sicuri il lavoro e la vita di chi lavora c'è, perché è proprio dal lavoro sicuro, dal lavoro in sicurezza, che deve prendere avvio ogni iniziativa economica. *(Applausi)*.

siamo ormai abituati all'atteggiamento di questo Governo che chiude le stalle quando i buoi sono ormai scappati e si ritrova sempre a inseguire gli eventi, come ha fatto con i provvedimenti sui *rave party,* con il decreto-legge Caivano e anche con questo provvedimento solo di facciata, per risolvere qualcosa, ma alla fine non risolve niente. Le uniche norme che riuscite a tirar fuori dal cilindro sono

sul vero tema che dovremmo affrontare: la prevenzione. *(Applausi)*. Questo è proprio un termine che non vi piace. Non riuscite proprio ad abituarvi all'idea che, se agiamo prima, non dobbiamo rammaricarci dopo, quando gli incidenti accadono. Questo provvedimento che avete varato in fretta e furia non fa altro che attuare una repressione dopo. Anche sulla patente a punti avete sprecato un'occasione, perché anche in i punti si perdono dopo, quando gli incidenti sono avvenuti, quando i morti ci sono stati. Addirittura un morto costa venti punti, come quelli della patente di guida. Dopo, per rimediare, un corso di formazione. Utile, peccato che le norme da oggi, anzi già da ieri, prima che varaste questo decreto, prevedevano che la formazione per i datori di lavoro dovesse essere norma di legge già dal 2022 e invece ancora aspettiamo il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni su questo. *(Applausi)*. Quando formiamo i datori di lavoro affinché capiscano che quello che investono nella sicurezza dei propri dipendenti è un valore aggiunto per le proprie imprese? Anche per i lavoratori autonomi la formazione è facoltativa - complimenti - nel mondo in cui viviamo di esternalizzazioni, un mondo in cui si fanno subappalti a cascata e poi magari l'ultimo anello della catena è quello più fragile, dove il lavoratore autonomo non è neanche obbligato ad essere formato sulla sicurezza. Neanche su questo siete intervenuti con questo provvedimento. Le poche cose che si potevano fare erano provvedere a una formazione preventiva, rafforzare la formazione nelle scuole e anche in tal senso dei provvedimenti sono in discussione alla Camera; ma anche quelli li avete talmente alleggeriti che diventano inutili, proprio perché prevenire, formare, educare sono concetti a voi estranei. L'unica cosa che conoscete è reprimere, aumentare le pene, ma mai niente che possa agire prima per salvare quelle vite, e non dopo che le abbiamo perse. *(Applausi)*. Lei si è vantata anche in quest'Aula, oggi, come in altre occasioni, delle assunzioni all'Ispettorato del lavoro: 1.700 unità, ma 1.000 di esse arrivano dalla scorsa legislatura per merito anche del MoVimento 5 Stelle. Quindi, come in altre occasioni, vi fate belli delle cose previste da chi c'era prima di voi. Ministra, agiamo in prevenzione, agiamo per salvare le vite, agiamo per formare chi deve avere la cultura della prevenzione e deve capire che ogni azione che compie può mettere in gioco la vita dei propri dipendenti. Cerchiamo di sollecitare il provvedimento alla Conferenza Stato-Regioni per la formazione dei datori di lavoro. Cerchiamo di dare un *imprinting* maggiore alla formazione dei nostri giovani sulla sicurezza. Se non cambiamo la mentalità sulla sicurezza fin da giovani, saremo sempre in quest'Aula a piangere qualche morto che bianco non è. Signor Presidente, ministro Calderone, colleghi senatori e senatrici, non si può morire per il lavoro, non si può uscire di casa e non ritornare più per un incidente sul lavoro nel 2024. Eppure, siamo ancora qui, dopo l'incidente di Brandizzo, dopo l'approvazione in quest'Aula della mozione votata all'unanimità, dopo varie tragiche morti ogni giorno - almeno tre, secondo le statistiche - e dopo la tragedia di Firenze. Nel primo mese del 2024 sono già 45 le vittime rispetto allo stesso mese del 2023, due in più. Non sono numeri, non sono statistiche, ma sono volti di persone, padri, madri, figli e figlie. Sono tragedie che colpiscono le famiglie. L'esternalizzazione del lavoro e dei servizi in appalti e subappalti è pericolosa, perché permette di ridurre al minimo la responsabilità, che viene così distribuita tra una miriade di soggetti, rendendo più difficile la comunicazione interna. Al tempo stesso, i ritmi diventano insostenibili. I contratti a termine sono un cappio al collo che obbliga a rispettare determinati tempi. Questo risponde alla logica egemone di massimizzare l'efficienza aumentando i profitti, riducendo i costi a discapito dei diritti dei lavoratori e delle loro sicurezza fisica ed economica. Ne va della loro dignità. Per questo bisogna contrastare la molteplicità delle forme di lavoro irregolare e soprattutto vietare i contratti pirata o quelli che vengono applicati sebbene la mansione che la persona viene chiamata a svolgere non sia quella coperta dal contratto che ha sottoscritto. Per esempio, agli interventi che hanno una prevalente connotazione edile deve essere applicato uno dei contratti dell'edilizia sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il contratto dell'edilizia più di ogni altro prevede un sistema strutturato e territorialmente diffuso in materia di sicurezza e formazione; per non parlare del contratto alle cooperative spurie, che applicano condizioni contrattuali illecite e sono le stesse cooperative regolari che ci chiedono di intervenire. Ci vuole più responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti: committente privato, appaltatore principale, subappaltatore, lavoratori. Spesso gli incidenti sono conseguenza di lacune progettuali, della mancanza di coordinamento delle lavorazioni, di tempistiche incompatibili con la natura e la complessità degli interventi. Proprio la rincorsa esasperata all'ultimazione delle opere costituisce frequentemente una criticità degli infortuni. Occorre una *governance* negli appalti sia privati che pubblici, prevalentemente in situazioni complesse, ma ugualmente indispensabile anche nei piccoli appalti per evitare interferenze anche a livelli inferiori. Solo attraverso l'utilizzo di organizzate procedure si garantiscono efficienza ed efficacia del sistema. Come Commissione monocamerale sulla sicurezza sul lavoro stiamo portando avanti la nostra analisi e, oltre alla *governance*, è stato rilevato che la condotta umana non risulta mai causa esclusiva e principale dell'infortunio. Essa è piuttosto una concausa che trova spesso la propria origine nell'assenza in capo al lavoratore di un'adeguata formazione, anzi di una cultura della sicurezza. Manca un'acquisizione di consapevolezza da parte del lavoratore che possa individuare in autonomia il rischio e prevenirlo. Riteniamo quindi importante la divulgazione della cultura nella sicurezza sul lavoro a partire dalle scuole- come state facendo - in coordinamento con il Ministero dell'istruzione e del merito e il ministro Valditara. In conclusione, la sicurezza sul lavoro dovrebbe essere intesa non solo quale obbligo imposto da una disciplina normativa, ma anche quale condizione di un diffuso benessere che si propaga e si esplica in tutti i suoi aspetti positivi, nei confronti di tutti i soggetti del sistema. bene aumentare le forze degli ispettori sul lavoro, fare in modo di semplificare e sburocratizzare il loro lavoro per essere presenti e attivi non solo come sanzionatori, ma anche come formatori e controllori. ottima la possibilità dei bandi di concorso regionali, che la Lega chiede da tempo su tutti i tipi di concorsi pubblici, per evitare sempre più vincitori che rinunciano a causa della lontananza delle sedi. In conclusione, Presidente, ringrazio il ministro Calderone, il ministro Valditara e tutto il Governo per le attività che sono già state messe in piedi finora e che lei, Ministro, ci ha illustrato. Sicuramente deve essere fatto un lavoro collaborativo tra le due Commissioni monocamerali del Parlamento e il Governo per poter arrivare a ulteriori soluzioni efficaci ed efficienti per garantire la sicurezza sul lavoro.

Sia io che lei veniamo non dalla politica, ma da esperienze sociali di rappresentanza del lavoro: io dei lavoratori, lei forse più da una rappresentanza vicino alle imprese, ma parliamo comunque di lavoro.

Quando parliamo di sicurezza, parliamo della priorità assoluta per tutti. Non c'è una parte che ha come priorità la sicurezza, perché parliamo del diritto alla vita delle persone. Ce lo dicono i dati che solo nell'ultimo anno ci forniscono una fotografia drammatica, e non solo per le oltre mille vittime del lavoro, ma anche per i 580.000 infortuni. ricordiamo poco perché sono tanti i morti che gli infortuni, alle volte gravi e gravissimi, sembrano quasi nulla. È un bollettino di guerra che abbiamo costantemente ogni giorno. Dietro a questi numeri ci sono tante vite rubate. Si muore male per lavoro; si muore ustionati, schiacciati, tritati. Così si muore per lavoro. E si lasciano sole famiglie disperate e bambini orfani. È una sconfitta per l'umanità non solo nel nostro Paese, ma in modo particolare nel nostro Paese.

ma su questo tema abbiamo un'occasione straordinaria, tutti insieme, di poter davvero finalmente scegliere una strada incisiva, reale, praticabile, che permetta di salvare tante vite. Mancano alcuni aspetti fondamentali, a partire da come si è trasformato il concetto della patente: prima i punti, ora i crediti. Non è soltanto una definizione diversa rispetto a come era originariamente. Le do atto che dal 2008 lei è la prima che ci mette le mani, ma bisogna mettercele bene. La trasformazione non è di poco conto. Non si tratta minimamente del tema di come cancellare la precarietà, uno dei fattori fondamentali per la sicurezza. Più avremo, in modo particolare in alcuni settori, lavoratori e lavoratrici precari, più morti continueremo a piangere. Non c'è nulla sull'eliminazione degli appalti a cascata. *(Applausi)*. Lo dico ai miei colleghi, anche a quelli che hanno sostenuto questo strumento: di appalto in appalto, da subappalto in subappalto, ci scappa il morto. È così. Prendete i numeri e le statistiche; se non volete, guardate le fotografie delle persone. Queste inquietano di più, ma già i numeri ci fanno capire, con grande chiarezza, che su tale materia va operato un cambiamento. Signora Ministra, facciamo insieme questa battaglia, per fare in modo che eliminare gli appalti a cascata aiuti a preservare la vita delle persone. Sì, c'è il rispetto dei contratti nazionali: ci mancherebbe. Ma questa dicitura che ogni tanto compare compare non è una differenza lessicale: è una differenza di riconoscimento della rappresentanza

davanti alle organizzazioni sindacali, quando è stato già fatto? Non era meglio discutere insieme di questi temi e insieme individuare quelle priorità che ci permettono davvero di essere incisivi? Poi ci sono delle cose che, onestamente, signora Ministra, proprio non capisco. In agricoltura, uno dei settori purtroppo più colpiti, in modo particolare

Lei ha parlato di come rafforzare i controlli. Io, pur essendo genovese, sono stata eletta in una splendida città del Sud, Palermo. A Palermo abbiamo tre ispettori del lavoro: che cosa vogliamo che controllino? Ci sono le assunzioni? Signora Ministra, per carità, meglio poco che niente, ma in questo caso il detto non è efficace. Sono

Aumentiamo il numero di assunzioni! Vale per gli ispettori come per le altre figure dell'Ispettorato. La patente a punti, quest'ultimo aspetto...

sicuramente, la necessità improrogabile di arrestare questo fenomeno che ci sconvolge ogni volta. Gli interventi che mi hanno preceduto mi hanno lasciato perplessa. Molti di quelli che sono intervenuti sembrano non aver vissuto in questa Nazione e soprattutto non aver in essa governato negli ultimi vent'anni. e lo ribadisco, indipendentemente dalle affermazioni di qualcuno, a cui voglio dire che i *rave* non si fanno più e che finalmente a Caivano c'è un po' di legalità ha attenzionato il problema della sicurezza sui luoghi di lavoro da subito, consapevole che le azioni da mettere in campo sono molteplici, ma conscio che *in primis* sia necessario mettere al centro il valore della sicurezza - come ha detto bene lei, Ministro - ovvero che si acquisisca e si promuova la consapevolezza su un tema a livello non solo sociale, ma anche individuale e, soprattutto, culturale;

in quelle scuole dove si apprende il concetto di diritti e doveri, e sottolineo doveri. Come diceva prima lei, Ministro, gli studenti di oggi saranno i lavoratori di domani, consapevoli di quanto il loro operare in ambito lavorativo possa incidere non solo su se stessi, ma anche sui loro colleghi. La formazione, quindi, deve essere alimentata continuamente; una formazione su misura, capillare, non formale, come spesso è avvenuto in questi anni, di cui forse tutti ci siamo dimenticati, ma sostanziale; una formazione adeguata che deve essere accompagnata dalla prevenzione e dal controllo; sì, quel controllo che va garantito da tecnici ispettori, grazie alle assunzioni che non sono avvenute con il Governo giallorosso

avviene anche attraverso l'introduzione della lista di conformità dell'Ispettorato nazionale del lavoro per i soggetti che dimostrino comportamenti corretti e rispettosi delle regole: una sorta di bollino blu che faciliti la scelta dei *partner* più affidabili negli appalti. Finalmente, da ottobre 2024, dopo sedici anni dall'introduzione del testo unico n. 81 del 2008, quello che tutti conoscete come testo sulla sicurezza, si passerà attraverso una patente a crediti (non a punti, ma a crediti), ovvero un titolo obbligatorio il cui possesso abiliterà imprese e lavoratori autonomi a operare nei cantieri. È una risposta dopo anni che, invece di incassare il plauso di tutte le parti sociali com'era accaduto quando la proposta proveniva dal Governo di centrosinistra, e non dimentichiamo che la propose nel 2021 il ministro Orlando - Orlando - oggi crea molti mal di pancia. Stamattina sui quotidiani il segretario della UIL la definisce indegna e il segretario della CGIL l'appella come strumento totalmente inadeguato e insufficiente. Non Non si riesce a capire cosa sia accaduto da allora, quando era il loro cavallo di battaglia. Non è cambiato molto in termini di fortuna. Ma c'è una differenza: al Governo ci siamo noi, noi che abbiamo il coraggio delle nostre azioni *(Applausi)*, credendo che questo sia uno strumento - come appena evidenziato - basato proprio sulla prevenzione e formazione; uno strumento di sicurezza conservativa e non punitiva che prevede decurtazioni in caso di illecito - ma abilita al riacquisto dei crediti attraverso l'implementazione della formazione; formazione - lo dico per un collega che mi ha preceduto - che non può essere diversa per i lavoratori di aziende di tre dipendenti rispetto ai lavoratori che ne hanno 1.000. La formazione è formazione e deve essere adeguata per tutti. uno strumento che, pur garantista, proprio come sancito dalla nostra Costituzione, consente, nelle ipotesi di infortuni più gravi, di sospendere in via cautelativa la patente sino a dodici mesi. Sì formazione, sì prevenzione, ma è anche necessario l'inasprimento delle sanzioni amministrative e penali di contrasto al fenomeno della somministrazione abusiva, dei distacchi illeciti e degli appalti fittizi; vale a dire di quei fenomeni patologici di decentramento produttivo in cui può annidarsi l'abbassamento delle soglie di sicurezza. Noi non abbasseremo mai la guardia verso queste forme illecite e patologiche che tolgono dignità al lavoro e dove la soglia di sicurezza non viene mai, - sottolineo mai - garantita. passi avanti importanti. È sicuramente necessario camminare insieme - e noi ci siamo - intervenendo in modo sistematico, coordinato su tutti gli strumenti utili al lavoro sicuro. Consapevolezza, formazione, prevenzione, conservazione e punizione, al fine di radicare nella coscienza individuale e sociale la cultura della sicurezza del lavoro.

alle quali risponderanno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso.

fanno emergere la necessità di interventi immediati e innovativi sul tema della sicurezza stradale. Lei già in questo senso sta promuovendo una serie di misure volte ad affrontare in modo organico la questione. Anche secondo gli ultimi dati pubblicati dalle associazioni, nel 2024 in Italia ci sono stati 350 morti e 280 feriti gravi, con un *trend* che non sembra tra questi un dato di rilievo riguarda i pedoni: da inizio anno ne sono morti 84 e la più alta incidenza di morti si riscontra proprio sulle strisce pedonali.

troppo poco incisive nel tutelare gli utenti più vulnerabili della strada. Fondamentale è anche il tema della ciclabilità. In molti Comuni le piste ciclabili sono state realizzate in zone altamente pericolose e spesso non sono accompagnate da una conforme segnaletica, creando delle difficoltà difficoltà sia per i ciclisti, ma anche per gli automobilisti e per la Polizia municipale. Quindi occorre un approccio alla cosiddetta mobilità dolce che sia pragmatica e che tenga conto della situazione in cui attualmente versano le strade del nostro Paese. All'interno dei centri abitati è infine necessario intervenire sulla diffusione incontrollata dei dispositivi di micromobilità elettrica, che costituiscono un ulteriore elemento di pericolo e che andrebbero ulteriormente regolamentati al fine di frenare il vertiginoso aumento di incidenti in cui sono coinvolti. Le chiediamo pertanto di sapere se e quali iniziative

precisare che il nuovo codice della strada è il risultato di un lavoro che dura da mesi, che ha coinvolto più di 100 realtà associative di settore che hanno trasmesso più di 200 contributi un quarto dei quali è stato recepito nel testo, che è poi stato affidato al dibattito parlamentare che in oltre sei mesi si è confrontato sul disegno di legge, abbinato ad altre proposte. Sono stati considerati 760 emendamenti, 70 modifiche e 94 ordini del giorno che rimarranno da esaminare la settimana prossima. Penso, quindi, che nessuno, se non strumentalmente, possa accusarci di aver fatto le cose in fretta o sulla base di posizioni non condivise con tutti i soggetti che si occupano di sicurezza stradale. Nel merito, parto da una questione fondamentale: il disegno di legge intende promuovere la sicurezza stradale intervenendo sia sulle sanzioni che sulla prevenzione. A quest'ultimo riguardo, si parla dell'educazione stradale vera sui banchi di scuola. Rispetto alle sanzioni, ricordo, fra le altre cose, la tolleranza zero nei confronti di chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe o ecceduto nell'utilizzo di alcol; ricordo l'aggravamento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida, visto che la prima causa di mortalità alla guida è, ahimè, la distrazione; ricordo la sospensione breve della patente di guida per diverse sanzioni, compreso l'abbandono degli animali lungo gli assi stradali. Sul piano della prevenzione, è prevista la tutela dei vulnerabili, ci sono piste ciclabili dedicate alle biciclette e non solo strisce di bianco tirate sull'asfalto. Si interviene sui monopattini con obbligo di contrassegno, casco e assicurazione; si interviene a tutela dei motociclisti con i *guardrail* salvavita, su cui stiamo investendo decine di milioni di euro. *ad hoc* finanziando 14 grandi Comuni per programmi per la sicurezza stradale riferiti ai pedoni, come l'interrogante richiamava. Stiamo lavorando con la Conferenza Stato-città ed autonomie per l'installazione di dispositivi di protezione per gli utenti deboli, comprese le due ruote. La sicurezza, quindi, da genitore prima ancora che da Ministro, è all'attenzione del Ministero e dell'intera

poco hanno a che fare con la sicurezza stradale. Quindi buon senso e concretezza senza ideologia. il Ministro per la sua puntuale e, come sempre, sollecita e dettagliata risposta. Alla luce di queste sue considerazioni, non comprendiamo le polemiche nate proprio di recente su una serie di norme volute dal Ministro

un'importante e - ne siamo convinti - decisivo passo in avanti sul piano della sicurezza. È quindi fondamentale che il nuovo codice della strada, dal Ministro fortemente voluto, possa entrare finalmente e pienamente a regime con l'applicazione anche ferrea delle tante norme che il Governo ha voluto introdurre, tenendo come faro la sicurezza non solo di chi è alla guida dei veicoli, ma di chiunque si trovi sulla strada, compresi quindi i pedoni, i ciclisti, gli utilizzatori dei monopattini. Anzi, siamo proprio certi che la nuova disciplina che regolamenta l'uso dei dispositivi di micromobilità elettrica svolgerà un ruolo chiave per ridurre gli incidenti e salvare vite. Ciò che serve è proprio il rispetto

come ha già detto il Ministro, con una grande attenzione alla formazione, che è fondamentale, perché il primo ambito sul quale si deve agire è proprio e soprattutto un cambio culturale, un cambio di mentalità che consenta davvero di far capire a tutti, ma soprattutto ai più giovani,

degrado in ogni luogo. Poi, sceso dal treno, dopo questa odissea, va a cercare un taxi e non lo trova, non ce n'è nemmeno uno, perché naturalmente questo Governo non solo difende i taxi, ma cerca di cancellare la possibilità da parte dei noleggi con conducente di fare il loro lavoro. quindi, una situazione di emergenza assoluta. Ebbene, di fronte a tutto ciò, ci si sarebbe aspettati, da parte del Governo, dei provvedimenti magari per mettere in discussione i vertici di Ferrovie dello Stato e di Trenitalia che non funzionano e si consente a questi vertici di fare cose allucinanti, come organizzare un treno ad alta velocità in Liguria per portare i giornalisti Rai al Festival di Sanremo o far fermare un treno perché il ministro Lollobrigida è in ritardo per andare a un'iniziativa, o provare a mettere in campo un provvedimento assurdo per limitare l'utilizzo dei bagagli, salvo poi ritirarlo il giorno stesso perché è una cosa ridicola, senza alcun senso. Ecco quello che sta succedendo nel nostro Paese. C'è poi il dramma più generale, quello che riguarda il futuro: cancellazione di opere previste dal PNRR (tratti della Palermo-Catania, tratti della Napoli-Bari,

organizziate ad ogni piè sospinto una finta inaugurazione per provare a mettere la polvere sotto il tappeto). Questa è la realtà. Lei è quello della legalità, quello che doveva sistemare il Paese e mi sarei aspettata, da una destra che non ha diminuito le tasse,

assolutamente diversi rispetto a quelli da lei riportati, per fortuna di chi utilizza quotidianamente il servizio pubblico. I dati di RFI aggiornati alla settimana scorsa per i servizi regionali parlano di una puntualità del 90,8 per cento; si può sempre far meglio.

Napoli-Bari e Terzo valico dei Giovi, l'obiettivo è di concludere i lavori come previsto entro il 30 giugno 2026. Quali siano le fonti di finanziamento ai pendolari interessa poco, a loro interessa semplicemente avere linee funzionanti. Le altre opere finanziate dal PNRR procedono tutte in linea con i traguardi del Piano e con la rimodulazione di dicembre abbiamo in aggiunta previsto un potenziamento del parco ferroviario per servizio Intercity con 13 ulteriori treni bimodali rispetto ai 53 già previsti e 30 ulteriori carrozze notte. Ricordo che l'80 per cento dell'utenza viaggia su Intercity, treni regionali e locali. Domani sarò nel pomeriggio a Reggio Calabria a presentare alcuni di questi nuovi Intercity. Concreti e tangibili sono gli interventi per rafforzare anche la sicurezza a bordo dei treni e all'interno delle stazioni, di nostra competenza. Ricordo i 1.000 militari in più

che arriveranno a una dotazione di organico di 1.500 persone che quotidianamente, soprattutto sulle linee più critiche, a rischio della propria sicurezza, garantiscono l'incolumità di lavoratori e passeggeri. In conclusione sulla questione taxi e NCC, che lei ha giustamente richiamato, irrisolta da sei anni e da tutti i precedenti Ministri, da mesi stiamo lavorando per recuperare il ritardo che - ripeto - risale a sei anni fa. Nel nostro Paese, ad esempio, non esiste un dato certo sul numero di vettori taxi e NCC perché nessuno ha avuto il coraggio di andare avanti su scelte amministrative di buon senso, come il registro informatico nazionale degli operatori del settore.

ad aiutare l'una o l'altra categoria, ma piuttosto a creare ulteriori possibilità di lavoro sia per i taxisti che per gli NCC, recuperando - ripeto - i sei anni, di chi mi ha preceduto, di zero al quoto.

alla guida di questo Ministero, come lei sa perfettamente. Potevate fare qualche cosa. Ciò che mi interessa della sua risposta è la negazione della realtà.

udite udite, non ci sono problemi ai taxi, udite udite, i treni sono puliti, udite udite, e va tutto bene, madama la marchesa. È cambiato il tempo in cui lei riusciva a raccogliere un po' di consenso da parte degli italiani perché magari raccontava delle cose che erano in sintonia con quello che il Paese davvero viveva. I lavoratori a cui lei si richiama, quelli verso i quali lei mi dice io devo portare rispetto, sono anche quelli che prendono i treni tutti i giorni e magari devono prenderli prenderli per andarsi a curare o per andare a lavorare in una fabbrica vicina, e si ritrovano a viaggiare in condizioni disperate perché lei non è in grado di realizzare le infrastrutture che sono tutte in ritardo, perché lei non è in grado di garantire i soldi del PNRR. Soprattutto però, Ministro, mi ha stupito che lei non abbia detto una parola quando il ministro Lollobrigida ha fermato quel treno, dimostrando un'arroganza incredibile nei confronti degli italiani, e quando Ferrovie ha organizzato un treno di alta velocità - beffa in Liguria, dove non c'è mai stata l'alta velocità - per portare i giornalisti Rai. Sa perché lei non l'ha fatto? Perché lei è un anello debole di questo Governo. Non c'è soltanto il fatto di non riuscire a realizzare le cose, c'è anche il fatto di non riuscire a farsi rispettare dentro questo Governo. Io vedo un'unica possibilità; se lei non è in grado di farsi rispettare, se non è in grado di realizzare, può fare sempre una cosa: dimettersi.

Signor Presidente, il ministro Salvini sa che, se c'è una questione che più fotografa il divario tra Nord e Sud è quella dei collegamenti ferroviari. Mentre, per andare da Roma a Milano, ci vogliono meno di tre ore, non è lo stesso per la Puglia. E dallo scorso 12 marzo, per raggiungere Bari, se va bene ce ne vogliono quasi sette Il drammatico aggravamento, in una situazione già difficile, come ben sa il Ministro, è per via della frana del tratto ferroviario tra Ariano Irpino e Montecalvo, che ha portato all'interruzione dei treni tra Foggia e Benevento. Rete ferroviaria italiana ha detto che i lavori per il ripristino richiederanno trenta giorni, sempre che non emergano ulteriori complicazioni legate alla particolare complessità dell'intervento. Subito dopo l'interruzione del tratto, è sopraggiunto l'immancabile aumento dei prezzi dei biglietti aerei, cosa che ha spinto il Codacons a presentare un esposto all'Antitrust. Un volo tra Brindisi e Roma è arrivato a costare fino a 750 euro, ma rincari importanti si registrano anche sui percorsi ferroviari alternativi. Per un biglietto del treno tra Bari e Milano si spendono anche 305 euro. Ad aggravare ulteriormente il quadro, la prevista interruzione anche di un tratto della linea adriatica, per lavori di ammodernamento che sono stati già programmati da Rete ferroviaria italiana. Mi auguro che quest'ultimo intervento venga posticipato alla fine dell'emergenza sulla tratta interessata dalla frana. Altrimenti, assisteremmo all'isolamento ferroviario della Puglia. In treno per la Puglia viaggiano professionisti, malati, studenti fuorisede ed un gran numero di turisti, anche stranieri. Si calcola che, tra Pasqua i turisti che intendono raggiungere la Puglia in treno siano oltre 80.000. Signor Ministro, si chiede allora di sapere se la tempistica prevista per il ripristino della linea Benevento-Foggia sia realistica, tenuto conto della situazione di elevato rischio idrogeologico che sta emergendo e quali interventi si intende predisporre sulla mobilità alternativa, a partire dal potenziamento dei collegamenti sostitutivi nella tratta tra Foggia e Benevento, per garantire piena mobilità da e verso la Puglia. Si chiede inoltre di sapere, quali iniziative urgenti si vogliono assumere per far fronte all'aumento dei costi, in particolare per calmierare l'incremento delle tariffe praticate dalle compagnie aeree e sui collegamenti ferroviari alternativi. Infine, quando e come saranno gestiti i lavori sulla tratta adriatica. ringrazio il senatore interrogante, perché mi permette di dare informazioni importanti, a lei e a tutti gli utenti della tratta dopo la frana all'interno della galleria Starza, lungo la linea Foggia-Napoli. Ho sentito i vertici di RFI pochi minuti fa, prima di venire in Aula. in Aula. Potranno essere più precisi martedì prossimo, dopo i primi versamenti di cemento, ma l'obiettivo è di finire in anticipo i lavori rispetto al previsto: quindi, entro la prima metà

degli utenti. In merito alle soluzioni di mobilità alternative al trasporto ferroviario, abbiamo lavorato fin da subito con Ferrovie dello Stato, che ha riprogrammato i servizi a lunga percorrenza, predisponendo anche un piano di collegamenti sostitutivi e di autobus. Ho chiesto, inoltre, che si possa sempre migliorare la qualità degli autobus sostitutivi, perché, onestamente, non è sempre all'altezza. Quindi, ho sensibilizzato Trenitalia affinché verifichi l'adeguatezza del programma di riprotezione

Abbiamo invitato la direzione competente del Ministero ed ENAC a monitorare l'attività degli operatori del trasporto aereo, per verificare l'applicazione di pratiche commerciali eventualmente scorrette. Alla luce di quanto accaduto, anche il Ministero dell'impresa e del *made in Italy* ha comunicato di aver esteso il monitoraggio dei prezzi delle tratte Roma-Bari, Milano-Bari, Roma-Brindisi e Milano-Brindisi nei periodi di interesse, in quanto originariamente non previste. In chiusura, doverosamente ricordo che, con la rimodulazione del PNRR, le risorse relative ai collegamenti ferroviari sono aumentate di miliardi di euro, come ho avuto modo di ricordare nella risposta precedente. Quanto agli interventi emergenziali sul dissesto idrogeologico, ricordo anche che i Presidenti di Regione tutti - sono commissari per la materia, come previsto dall'ordinamento vigente. Il Governo è ovviamente al fianco degli enti territoriali per supportarli negli interventi che devono eseguire. In queste ore sono in contatto con il sindaco di Lovere, nell'alta Lombardia per una frana e con il sindaco di Maratea per la riattivazione della strada in tempi utili per la stagione turistica. Ovviamente sono eventi che non si possono prevedere: quello che è nostro onore e onere fare è garantire un servizio sostitutivo all'altezza e tempi certi per la riattivazione delle linee. La ringrazio e spero di avere notizie ancora migliori a metà della prossima

c'è: è vero che ci sono gli autobus sostitutivi, ma non è stata comunicata l'esistenza degli stessi, per cui chi sta cercando quel treno a lunga percorrenza non ha le indicazioni,

Allora forse non c'è solo il problema di intervenire celermente nel momento in cui ci sono frane, ma c'è il problema di chiedersi se non sia necessario fare dei seri lavori infrastrutturali di tutela, visto anche il cambiamento climatico, che lei spesso nega, Ministro, e che invece ci attraversa, e cominciare a dire che l'investimento infrastrutturale nel Mezzogiorno deve essere davvero considerato una priorità del Governo. Governo. Così però non è. Il problema non è dire ai cittadini qual è la fonte del finanziamento in un caso o nell'altro; la questione è che continuiamo ad avere un servizio ferroviario tutto spostato sul Nord, in parte sull'asse adriatico, ma che non collega il Mezzogiorno,

per Bari e farlo rapidamente, oltre a mettere in funzione i tratti ferroviari in Sicilia, che non ci sono, e a rendere possibile la vita quotidiana delle persone che hanno bisogno dei treni e spesso non li trovano.

ministro Sangiuliano, come lei sa molto bene, il Piemonte è un territorio ricco di luoghi di cultura che attirano turisti da tutto il mondo, comprendendo ben quattro siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tra questi le Residenze sabaude, un complesso costituito da 22 palazzi e ville di grande pregio storico ed architettonico, la metà delle quali situate nella città di Torino e l'altra metà realizzate con una pianificazione radiale intorno alla città fra il XVI e il XVII secolo, cioè uno straordinario esempio di pianificazione urbanistica e di costruzione di un'architettura monumentale iniziata da Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dopo il trasferimento della capitale del ducato a Torino nel 1562, realizzate dai maggiori architetti e artisti dell'epoca. Ebbene, nel 2023, il solo complesso della Reggia di Venaria, che ricordo circa vent'anni fa le giunte di sinistra volevano abbattere e fortunatamente, invece, ingenti investimenti hanno permesso di 2023 il solo complesso della reggia di Venaria ha registrato 446.000 visitatori, riuscendo ad abbinare mostre temporanee alle visite all'importante patrimonio culturale permanente della reggia, sede di grandi eventi. Basta ricordare che il prossimo 26 e 27 aprile si terrà presso la Reggia il G7 energia e ambiente. Purtroppo, però, le altre residenze sabaude non hanno il successo di visitatori della Reggia, anche se sono state restaurate e sono aperte al pubblico, anche se hanno da offrire molto dal punto di vista culturale. Penso a Palazzo Reale, a Palazzo Carignano, a Villa della Regina, alla Palazzina di caccia di Stupinigi e al Castello di Racconigi. Le chiediamo quindi, signor Ministro, quali sono le azioni che ha intrapreso e intende intraprendere per dare ulteriore valorizzazione alle residenze sabaude, soprattutto mettendole in rete, posto che sono inserite in un territorio unico, quello piemontese,

ringrazio, senatore Rosso, per questa interrogazione e le do subito una notizia: domani sarò a Venaria e questa mia presenza non era stata certo prevista sapendo della sua interrogazione, ma è stata concordata da molto tempo. Tra l'altro, non è la prima volta che mi reco da Ministro a Venaria, perché ne ho ben presente l'importanza storica, architettonica, artistica, di grande valore per tutta l'identità nazionale. il dettato dell'articolo 9 della Costituzione, che ci impone la valorizzazione di questa grande meraviglia, le do alcune informazioni: negli ultimi anni il Ministero della cultura ha destinato a Venaria oltre 127 milioni di euro è in corso di definizione un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro per vari interventi in palazzi, ville statali e non, che compongono appunto il sistema delle residenze reali. Domani annunceremo a Venaria l'arrivo della grande mostra di Capodimonte: la stessa che è stata esposta al Louvre a Parigi verrà esposta a Venaria, con opere di Tiziano, di Masaccio e altri grandissimi maestri. Ancora, le voglio dire che domani, ai Musei reali di Torino - anche se i Musei reali non appartengono a questo sistema - è prevista l'inaugurazione della mostra su Guercino. Le dico anche che i Musei reali di Torino sono stati da me portati in prima classe. Stranamente la città di Torino, il Piemonte, non aveva un museo di prima classe. Adesso ce l'ha nei Musei reali di Torino, cosa che io ritengo assolutamente doverosa. Inoltre, le dico che sempre ai Musei reali, il 27 marzo si inaugura la mostra «L'autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro», posta sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Regione Piemonte, con l'esposizione di oltre 60 opere. Ma noi abbiamo un tavolo permanente con il Presidente della Regione e con il sindaco di Torino, perché siamo consapevoli che bisogna intervenire in termini infrastrutturali,

ovviamente soddisfatto della sua risposta. Non ci siamo messi d'accordo sul fatto che lei venisse domani, però è testimonianza della vicinanza e dell'importanza che lei dà al patrimonio culturale torinese e piemontese. però possiamo fare un passo successivo e possiamo veramente andare a mettere in rete quelle residenze meno conosciute, i nostri gioielli culturali, con un approccio olistico, per poter ottenere successi che altri Paesi hanno ottenuto. Faccio un esempio: penso ai Castelli della Loira. Quando un turista li va a visitare, viene convinto, guidato, accompagnato a vederli tutti, attraverso la bigliettazione unica, le informazioni e le mappe presenti in tutti i siti. Un percorso che, senza accorgersene, diventa quasi obbligato. Sono sicuro, Ministro, che la nostra maggioranza e lei lavorerete sempre più efficientemente per mettere in rete le residenze sabaude, con l'obiettivo ulteriore di costruire un percorso sensoriale che si allarghi anche alle altre ricchezze culturali del Piemonte. un patrimonio che non è solo architettura e opere d'arte, ma anche una cultura di eccellenze artigiane (penso per esempio alle ceramiche di Castellamonte), ed una cultura enogastronomica (penso al vino, al tartufo d'Alba, alla tradizione culinaria). Mettere in rete tutte queste culture può essere una grande risorsa per il Piemonte, che purtroppo gradualmente esce da una vocazione industriale legata all'*automotive* e deve trovare altri percorsi di crescita. Quello legato al turismo culturale è uno di questi e rappresenta un *win-win*, perché da una parte crea ricchezza e lavoro sul territorio e dall'altra mette a disposizione di milioni di persone un'esperienza culturale e sensoriale indimenticabile.

Signora Presidente, signor Ministro, da troppo tempo ormai assistiamo alla progressiva chiusura e allo smantellamento di gran parte dei corpi di ballo stabili nelle fondazioni lirico-sinfoniche, disperdendo così un grande patrimonio artistico e culturale nazionale. Attualmente, come lei sa, signor Ministro, permangono attivi solamente quattro corpi di ballo stabili, ovvero Milano, Roma, Napoli e Palermo. Proprio per questo motivo il MoVimento 5 Stelle ha depositato - ed è attualmente incardinato in Commissione cultura al Senato - il disegno di legge n. 568, che ha tra gli obiettivi proprio quello dell'apertura di nuovi corpi di ballo stabili nelle fondazioni liriche, eventualmente anche con la modalità della condivisione tra due fondazioni. Il 19 marzo, ovvero pochi giorni fa, c'è stato un incontro al Ministero tra il sottosegretario Mazzi e vari operatori e lavoratori del settore. Al termine di questo incontro avete annunciato l'apertura di due nuovi corpi di ballo, uno in collaborazione tra le fondazioni di Verona, Venezia e Trieste, e un altro in collaborazione tra le fondazioni di Bologna e Firenze. La prima cosa che ci siamo domandati è perché escludere dal progetto città come Torino, Genova, Bari, Cagliari, visto che invece nel nostro disegno di legge prevediamo una modalità che coinvolgerebbe tutte le fondazioni liriche italiane; modalità questa che, a nostro avviso, dovrebbe essere considerata e perseguita. Vengo alle domande, signor Ministro. Le chiediamo quante risorse volete investire in questo progetto. Le chiediamo quali saranno le garanzie contrattuali dei ballerini professionisti, cioè di artisti che ci invidia tutto il mondo e che come tali vanno trattati. Saranno dei dipendenti a tempo indeterminato di una fondazione, che sarà quindi la loro effettiva sede di lavoro, o saranno dei precari a vita costretti a migrare di città in città ad ogni produzione? Avete intenzione di prevedere nel FUS, oggi Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV), dei requisiti per incentivare le fondazioni a realizzare produzioni di balletto con corpi di ballo stabili? Infine, signor Ministro, quali sarebbero i criteri per cui avete deciso l'esclusione delle fondazioni di diverse città da questo progetto? Perché a Firenze sì e a Torino no? Perché a Bologna sì e a Genova no? Quale sarebbe la logica? Non sarebbe forse meglio creare le condizioni per permettere a tutte le fondazioni liriche di poter disporre di un proprio corpo di ballo stabile, anche se in collaborazione con un'altra fondazione, così come prevede il nostro disegno di legge?

Gli altri hanno chiuso le fondazioni lirico-sinfoniche e i corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche. Ne sono rimaste soltanto quattro: il Massimo di Palermo, la Scala, il San Carlo, l'Opera di Roma. Noi intendiamo riaprirle. Proprio perché intendiamo riaprirle, vogliamo fare una politica di passi ponderati e saggi, quindi non promettere tutto a tutti, ma cominciare con una formula più elastica, più pratica, ossia quella di prevedere corpi di ballo che possano coprire più fondazioni: Venezia Venezia e Verona, che hanno una contiguità geografica; Firenze e Bologna, che pur essendo in Regioni diverse sono ben collegate. Nulla esclude che successivamente, negli anni a venire, possiamo allargare lo spettro e quindi coinvolgere ad esempio Genova. Del resto, lei è stato consigliere di amministrazione, anche in un macroscopico conflitto di interessi, della fondazione lirico-sinfonica di Genova. Non mi risulta che lei, da consigliere, abbia mai richiesto o segnalato la necessità di ricreare un corpo di ballo. Ha cambiato idea? Benissimo, le faccio i miei più vivi complimenti per aver aderito a quella che è la nostra posizione. Al tavolo del 19 marzo Noi stiamo pensando ad un provvedimento normativo in cui sancire la nascita di questi due nuovi corpi di ballo, che - glielo ripeto - non precludono in futuro alla creazione di corpi di ballo a Genova, a Torino, a Bari e ovunque lo si creda. Lo faremo con un provvedimento normativo e stiamo ipotizzando per il 2025 l'istituzione di un ulteriore fondo da assegnare previa presentazione di progetti di sviluppo delle attività pluriennali, secondo i criteri definiti con apposito decreto del Ministero. del Ministero. È ovvio che non dobbiamo creare alcuna forma di precariato. Ci atterremo scrupolosamente a quello che stabilisce il contratto di lavoro in questo ambito. I danzatori di questi nuovi di questi nuovi corpi di ballo saranno trattati come quelli del Teatro alla Scala, del Teatro San Carlo o del Teatro dell'Opera di Roma: avranno il medesimo trattamento e questo mi sembra abbastanza scontato. Noi stiamo dando grande attenzione alla danza, perché crediamo nell'espressività di questa forma di arte, che tra l'altro coinvolge - le do una notizia - tantissimi giovani. Sono tanti i giovani che oggi praticano la danza in Italia, ben venga, e siccome vogliamo cercare di offrire loro una prospettiva, magari una una visione su dove finalizzare questo loro impegno e questa loro attitudine culturale, stiamo operando con grande impegno. Tra l'altro, io personalmente ho nominato alla Presidenza del Consiglio superiore dello spettacolo Eleonora Abbagnato, che è un'eccellenza di questo settore.

Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la consueta polemica fuori luogo. *(Applausi)*. Le do una notizia: nelle fondazioni liriche italiane non ci sono i consigli d'amministrazione, ma i consigli di indirizzo. Glielo dico perché lei è il Ministro della cultura e dovrebbe saperlo. Abbiamo capito che lei legge poco e vota cose che non ha letto,

è che lei viene qua senza un testo di legge ma avendo già fatto un comunicato stampa; noi, invece, abbiamo depositato un disegno di legge. Lei capisce che parlare di fare un comunicato stampa su qualcosa che non esiste ancora, su un testo che non c'è, è come votare un libro che non si è letto, cioè è una cosa che veramente non ha senso, ma sappiamo che lei di questo è un esperto. Mi fa piacere la parte finale del suo intervento. Purtroppo lei ha questa aggressività repressa, che probabilmente ha a che fare con la sua adolescenza, con la sua infanzia. Non lo so, però sarebbe meglio che non portasse ogni volta questa aggressività in quest'Aula, invece si portano delle proposte, signor Ministro. Noi ne abbiamo fatte e infatti c'è un disegno di legge che riguarda questo tema. Aspettiamo un vostro testo per poterlo discutere e, invece di fare polemica inutile come lei fa ogni volta, poter dar dignità a quei lavoratori e a quegli artisti che non ne hanno e per i quali è importante che tutti insieme ci si metta a lavorare, per dar loro dignità e restituire anche quella qualità professionale che non possono avere. La polemica che lei fa ogni volta, mi creda, non è all'altezza del ruolo che ricopre.

chiede di riferire su alcune sue recenti dichiarazioni in merito all'ampliamento di sedi di alcuni grandi musei, quali gli Uffizi di Firenze, il Museo archeologico di Napoli e la Pinacoteca di Brera a Milano. Ovviamente l'ordine è solo casuale.

prevista dall'articolo 9, cioè la tutela e la conservazione come funzione primaria del suo Ministero, ma anche, ovviamente, la cultura come elevazione civica, intellettuale e spirituale.

e anche rispetto al PIL, le spese per la valorizzazione del patrimonio culturale sono molto inferiori. Quello che ci preoccupa, però, non è tanto il fatto che noi esponiamo solo più o meno il 10 per cento delle opere (480.000 dei cinque milioni di opere che abbiamo), quello che ci preoccupa è quello che abbiamo ereditato, quello che lei ha ereditato nel Ministero, ovvero un'assenza totale di consapevolezza del valore economico, oltre che umanistico, del nostro patrimonio culturale, in sostanza che la cultura non è solo un costo, ma una risorsa, come lei sta dimostrando con alcune sue recenti iniziative. Ne cito solo un paio: quella del Pantheon qui a Roma, che è stata un'iniziativa di grande successo, ma anche le nuove 17 autonomie museali che lei ha saputo ridelineare, proprio per mettere in chiaro che per noi la cultura non è solo conservazione, non è solo un costo, ma è anche valorizzazione, dal punto di vista sia delle entrate dirette, sia del grandissimo indotto che si può generare per il Paese. Per questo le le chiediamo di descriverci quello che lei ha delineato come ampliamento di queste tre grandi strutture museali, sapendo che non saranno né le prime, né le ultime nel suo mandato, iniziato da appena sedici mesi.

senatore interrogante per questa domanda che mi consente, appunto, di raccontare quello che stiamo facendo. Ho detto che intendo raddoppiare lo spazio espositivo e le strutture di tre grandi siti museali italiani. Il primo progetto posso annunciare che nel prossimo autunno apriremo palazzo Citterio, un edificio molto bello nel cuore di Brera, che fu acquistato nel 1972 dal Ministero della cultura e poi dopo, chissà per quale mistero, non si è riusciti mai a concretizzare il progetto. Ho dato personalmente impulso al progetto, recandomi sei volte all'interno di palazzo Citterio proprio per verificare l'andamento dei lavori e credo che finalmente in autunno potremo raddoppiare l'esposizione di Brera con questo edificio, dove troverà spazio tutta la collezione del Novecento. Lo stesso stiamo facendo per quello che forse è il più prestigioso museo italiano, il Museo degli Uffizi: addirittura lì gli spazi saranno triplicati, con due nuove strutture, le due ville medicee di Careggi e di Montelupo Fiorentino. Nel caso di Careggi, i lavori sono quasi conclusi e quindi lì troveranno spazio le collezioni degli Uffizi che al momento non vengono esposte. La terza tappa è Napoli, dove stiamo recuperando con i fondi del PNC l'ex Albergo dei poveri in Piazza Carlo III, monumentale edificio di 140.000 metri quadrati (per capirci, gli Uffizi si estendono per 90.000 metri quadrati) e lì raddoppieremo la presenza del Museo archeologico nazionale di Napoli, che è ritenuto uno dei più importanti musei archeologici al mondo, raccogliendo anche i tanti tesori che vengono dagli scavi che sono stati rifinanziati in legge di bilancio e che stiamo comunque portando avanti sia nell'area di Pompei, sia nell'area di Ercolano. Non ci fermiamo soltanto a queste tre tappe, però, perché sta per aprire a Firenze il Museo della lingua italiana, a Milano stiamo lavorando per avviare - la struttura è già stata individuata - il Museo dell'arte digitale e poi ci sono i due grandi progetti del Museo della Shoah a Roma, che è stato appunto varato con leggi approvate all'unanimità dal Parlamento, e il Museo del ricordo, sul quale c'è un disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri che fra poco approderà nelle Aule parlamentari.

soddisfatto della sua risposta. Essa è un pezzo di un mosaico che ci ha già fatto intravedere, che non tutela solo la memoria storica e l'identità culturale, ma anche la valorizzazione - perché no? - la scoperta di tutti quei talenti nascosti che sono nei magazzini dei nostri musei e la consapevolezza che questa valorizzazione sia un percorso affinché

Io non sono sempre un amante degli interventi di fine seduta, ma se uno si chiama come un calciatore dell'Inter, come faccio a negarglielo? Ne Signor Presidente, la comunità del Partito Democratico è stata colpita in questi giorni da due lutti non imprevisti, ma altrettanto dolorosi. Vorrei maledire la malattia implacabile che si è portata via in poco tempo due dirigenti del nostro partito, Maurizio Chiocchetti e, ieri, Lino Paganelli, con i quali ho avuto il privilegio di collaborare al Nazareno. qualcosa delle vite di questi uomini, delle sigarette di Lino o del suo sguardo di sottecchi, ma non spetta a me, che non sono stato compagno; pare sempre di abusare, di dire un indicibile che può essere soltanto ricordato e tramandato come un sussurro. C'è stato il tempo della rabbia e dell'amarezza accanto a quello delle grandi responsabilità per entrambi, per Maurizio e per Lino. La sua Festa dell'Unità, dove festa e unità erano due parole che Paganelli aveva cuore e che dovremmo avere a cuore tutti noi che di politica siamo fatti. La politica come festa e come unità. ieri mattina al funerale c'erano tutti; Elly, Walter, Nicola, anche quelli - e voglio rendere loro onore - che con Lino hanno lavorato e che oggi guidano o militano in un altro partito, tra i quali Maria Elena e Francesco. Vorrei però concludere in un "amaretto" personale recente il senso di queste parole qui al Senato per condividere con voi chi fossero questi uomini. Sono andato a trovare Lino Paganelli nella struttura dove era ricoverato qualche giorno fa, assieme al senatore Fina e alla segretaria del mio partito Elly Schlein. Era arrivato, stremato, con le mani strette nelle sue mani, Elly informava Lino delle ultime novità della campagna elettorale. Lui che era stato tra i più esperti nella balistica e nell'idraulica dell'organizzazione. Lino era sofferente e silenzioso, si addormentava ripetutamente, sembrava già altrove. Era Era bellissimo, anche tra quelle lenzuola, con i capelli nerissimi. Attorno la sua famiglia; lo splendido sorriso di Gaia e le persone che lo hanno amato. Un pensiero va a Gabriella. A un certo punto, Presidente, Elly gli ha detto quanto il partito dovesse a lui per il suo lavoro, per l'impegno che aveva messo in tutti questi anni. Improvvisamente, aprendo gli occhi che erano stati chiusi fino a quel momento, Lino le ha risposto chiaro e secco, con un estremo fulmine benevolo nello sguardo: no, Sono io che devo tutto al partito. Ecco, Presidente, sono sicuro che lei mi comprenderà, come uomo delle istituzioni e di partito. Vorrei che anche lei, come ognuno di noi in quest'Aula, sentisse la dignità e la forza che vibra in questo testamento. Possiamo scontrarci aspramente, lo facciamo quotidianamente, essere in disaccordo su tutto, polemizzare. Ci mancherebbe. La voce che arriva però a quest'Aula, se ce ne è una residua, non è solo quella che promana dal voto dei cittadini, ma quella di questo strumento che fu potente e oggi è esile e celibe, che sono i partiti, che sono fatti di rappresentanti e dirigenti, di funzionari e militanti, di volontari e di persone, come Maurizio, Lino e come Mario Giachini, scomparso qualche mese fa, delle loro famiglie e delle loro esistenze, che ci restituiscono il senso del decoro, del dovere e del rispetto che ognuno qui, oggi, in quest'Aula, vorrei che sentisse. Uomini di partito, del Partito Democratico in questo caso, e non solo di parte, di una comunità viva, talvolta feroce e distratta, ma viva. Concludo, Presidente, se avessi un cappello, me lo toglierei per Lino, se avessi ancora occhi, li chiuderei anche io, se avessi voce, ma è finita. *(Applausi)*.